Onorevoli colleghi, «Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Con questa affermazione si apre la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui ricorre oggi il 60° anniversario. Subito dopo, la Dichiarazione ricorda «che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità». La dichiarazione che oggi celebriamo non nasce dunque da un pensiero astratto, da un ideale assoluto, ma si radica nella tragica lezione della storia: l'offesa portata dal totalitarismo alla "coscienza dell'umanità". In questo clima l'Assemblea costituente approvò la nostra Carta fondamentale, di cui sempre quest'anno abbiamo celebrato il 60° anniversario. La nostra, come le altre Costituzioni del dopoguerra, si apre con il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, La nostra, come le altre Costituzioni europee del dopoguerra, fissa poi quel principio di apertura al diritto e alle organizzazioni internazionali che segna uno spartiacque fondamentale nella storia e nella natura stessa dei nostri Stati. La sovranità non equivale più a onnipotenza. Viene superata quella carica ideologica che aveva portato ai conflitti che hanno insanguinato il Novecento. Su queste fondamenta si è sviluppato il processo di integrazione europea che ha ricomposto il nostro continente, dilaniato nei secoli da guerre, in un unico spazio di sicurezza, libertà e giustizia. Oggi, celebrando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, una volta di più dobbiamo ricordare, specie ai più giovani, la forza e il valore di questi principi che costituiscono il fondamento della nostra convivenza, in Italia, in Europa e nel mondo. Con orgoglio dobbiamo rivendicare l'azione che il nostro Paese conduce nella comunità internazionale a favore della promozione e della tutela dei diritti umani, nella convinzione, così chiaramente scritta nella nostra Carta costituzionale, che il loro rispetto costituisce un valore essenziale e al contempo condizione indispensabile per garantire pace e giustizia. Dieci anni fa qui a Roma abbiamo ospitato la Conferenza che ha adottato lo Statuto della Corte penale internazionale; italiana è stata l'iniziativa della campagna per la moratoria della pena di morte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a tutela del diritto - quello alla vita - più sacro e inviolabile. Ed ho appreso con piacere dal neo Presidente della Commissione diritti umani, il collega Marcenaro, che la Commissione stessa inizierà i propri lavori proprio nella giornata odierna. Oggi, colleghi, di fronte a nuovi «atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità», alla cieca violenza del terrorismo, alle violenze che feriscono la libertà religiosa (e non posso non ricordare qui in Senato la mozione che poche settimane fa abbiamo insieme approvato sulle terribili violenze contro i Cristiani), dobbiamo ricordare una volta di più la scelta di valore che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite fece 60 anni fa, proclamando, come la più alta aspirazione dell'uomo, «l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno». Che questo possa avverarsi, in un mondo che ha il dovere di credere ancora nelle ragioni della speranza, è l'auspicio - ne sono certo - di tutto il Senato.

richiede di essere affrontata con spirito critico. Non voglio indulgere ad un approccio armonico perché sarebbe troppo facile. Penso sia più rispettoso dello spirito della Dichiarazione dei diritti dell'uomo considerare quanto essa sia stridente nei confronti della realtà internazionale e anche nazionale. Per quello che riguarda il profilo internazionale, basterebbe ricordare ciò che hanno scritto illustri giuristi statunitensi sul significato intimamente anticostituzionale del carcere di Guantanamo: la sospensione dei diritti costituzionali basata sull'arbitrio, sulla detenzione senza termini, sulla incertezza del destino futuro. Un tema che è stato sfiorato, ma che è stato poco approfondito. Per corrispettivo si potrebbe ricordare l'indifferenza pressoché generale nei confronti della violazione dei diritti umani in Russia, dove centinaia di giornalisti sono stati ammazzati quasi esclusivamente perché raccontavano una realtà scomoda. Quanto l'indifferenza nei confronti di questo fenomeno così abbietto sia generale l'ha testimoniato paradossalmente ad un certo punto anche il Presidente del Consiglio italiano, quando una giornalista ha fatto una domanda sull'assassinio di Anna Politkovskaja ed egli ha pensato di sottolineare il suo dissenso con un curioso gesto della mitraglietta. I diritti umani sono violati anche in Italia. Il tema della schiavitù, della tratta dei corpi

possiamo ascoltare con attenzione gli interventi dei senatori sull'argomento con il quale ho aperta questa seduta? Non credo sia un tema di secondaria importanza. Prego, senatore Pardi, e stavo giungendo a considerare la violazione dei diritti umani nella nostra terra. Lo spirito fondamentale di questa dichiarazione, infatti, è l'impegno autocritico: non si può pensare di affermare i diritti nel Grazie, situazione sociale italiana ci dice che in Italia i diritti umani sono spesso e costantemente violati, soprattutto per quanto riguarda la condizione di vita di coloro che vengono a lavorare in modo irregolare, senza senza permessi, privi di cittadinanza e sottoposti a una sorta di controllo stringente sulla loro vita, sui tempi di lavoro, sulle condizioni di esistenza.

che si è finto più volte emigrante e si è andato a cacciare in condizioni difficili nei centri di accoglienza temporanea, nei campi dove si raccolgono i pomodori, dove si svolge il lavoro agricolo senza protezione. inchieste testimoniano come la vita di decine di migliaia di persone, che fanno da tessuto connettivo di un lavoro senza nome e senza speranza, sia sottoposta a condizioni inenarrabili che che stanno davanti alla coscienza critica della Nazione come un memento di fronte a cui non bisogna mai voltare il capo.

della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Entrambe queste carte fondamentali sono seguite alla Seconda guerra mondiale e quindi hanno nello spirito e nel dettato tutto l'anelito al riscatto dell'umanità e al riconoscimento dei diritti fondamentali. Per parlare più direttamente della Dichiarazione dei diritti umani, firmata il 10 dicembre 1948, ricordiamo che si tratta di un codice etico, di un documento che per la prima volta nella storia dell'umanità ha fissato quali siano i diritti che toccano l'individuo. sue spalle, ovviamente, ci sono stati filosofi di fondamentale valore, e vale la pena di ricordare che Jacques Maritain partecipò di persona alla stesura del testo della dichiarazione. Così come vale la pena di ricordare la stagione dei diritti sanciti durante la Rivoluzione francese, accolti in questa carta un documento costruito in 30 articoli, ognuno dei quali, nella essenzialità dei suoi titoli, esprime principi profondi e universali. è una sorta di inno alla libertà in tutte le sue dimensioni ed espressioni, alla democrazia, al diritto alla vita, ma anche alla sicurezza della persona.

occorre dire che dinanzi a una carta di questa portata, collaudata in 60 anni, nei quali non sono certo mancati i conflitti, non si possono certo dimenticare i quotidiani soprusi che dittature fondamentaliste esercitano - in special modo sulle donne, trattate ancora come schiave - con crudeltà quando non con la tortura. È un bel ripasso, una bella lezione per tutti noi, guardare da vicino la Carta per scoprire il il diritto alla *privacy* e per riconoscere quel garantismo spesso dimenticato alla nostra latitudine. Che dire poi di quelle parti essenziali riguardanti la libertà di pensiero e di espressione, tanto care alla tradizione della Lega Nord, per non parlare della sicurezza alla quale ha diritto ogni individuo? In sostanza, ci troviamo di fronte ad un documento corposo, ancorché essenziale, che che allinea tutti i diritti fondamentali dell'uomo e li traduce in una sintesi che, purtroppo, è ancora ignorata in molte parti del mondo e, per qualche verso, riscontra dei vuoti anche nell'assetto sociale del nostro Paese.

e sappiano aprire nuove frontiere per un mondo più giusto, più libero e capace di prospettare per le future generazioni una qualità della vita che sappia coniugare sviluppo e progresso. Grazie, signor Presidente. Presidente, inizierò il mio intervento ricordando le due personalità che più di altre hanno contribuito alla stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il primo è René Cassin, insigne giurista francese. Ha combattuto, è stato ferito ed ha vissuto gli orrori della prima guerra mondiale; in seguito, ha assistito alla nascita e all'affermazione del fascismo e del nazismo, alla loro violenza, ed è stato il primo civile a rispondere all'appello per la Francia libera che Charles de Gaulle lanciò dai microfoni di Radio Londra. La seconda è Eleanor Roosevelt. È stata a fianco del marito, Franklin Delano Roosevelt, Presidente di un'America che ha dovuto affrontare, nel corso dei suoi mandati, la crisi economica e sociale più profonda e la minaccia più e la minaccia più grave alla vita e al futuro...

universale con il primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 si può notare un piccolo cambiamento: la parola "uomini"

oggi sono, in primo luogo, i diritti delle donne. I tre quinti delle persone più povere del mondo condannate alla fame e private del diritto alla vita sono donne e bambini. Sette su dieci dei bambini che non vanno a scuola sono bambine. Mezzo milione di donne muoiono ogni anno durante il parto e, se ciò non bastasse, ci sono ci sono i talebani a ricordarci che i nemici dei diritti umani sparano il loro primo colpo contro le donne. Se le donne saranno libere dalla violenza, se saranno in buona salute e riceveranno una buona educazione, se avranno la possibilità di lavorare e guadagnare come partner a pieno titolo e con pari diritto nella società, le loro famiglie fioriranno. E quando le famiglie fioriscono allo stesso modo fioriscono la comunità e la Nazione. «I diritti umani sono i diritti delle donne e i diritti delle donne sono i diritti umani». Queste parole le pronunciò Hillary Clinton, la donna che nel 1995 guidava la delegazione americana alla Conferenza mondiale di Pechino e che oggi è il nuovo Segretario di Stato americano. Esistono finalmente le condizioni internazionali per una nuova fase di lotta per i diritti umani, e mentre esprimiamo la soddisfazione per il successo della moratoria, non possiamo non vedere la ferocia delle impiccagioni pubbliche in Iran, non possiamo non ricordare l'assassinio di Anna Politkovskaja in Russia, non possiamo non vedere la repressione che nega al Tibet l'autonomia alla quale ha diritto. E credo che noi tutti dobbiamo un ringraziamento al presidente Sarkozy

siano scossi, minacciati, travolti dalle nuove guerre che insanguinano la terra, che talvolta assumono il carattere di veri e propri genocidi e che, in ogni caso, sempre più estesamente coinvolgono vittime civili. Questo sono oramai le guerre. Diritti umani, democrazia, Stato di diritto: sono termini difficili da separare. Ce lo ha ricordato un grande teorico, al quale è stato riconosciuto l'onore del premio Nobel, Amartya Sen. Noi vogliamo una politica estera italiana ed europea che abbia nei diritti umani un suo pilastro, una politica estera che in questo caso non riguarda solo le strutture della diplomazia, ma anche, nel mondo globale, le imprese e i loro comportamenti, la cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni non governative, cioè che richiede un impegno corale di un insieme di soggetti. Propongo, signor Presidente, e le chiedo di considerare questa possibilità, che anche come fatto simbolico il Senato valuti l'opportunità di istituire un premio per i diritti umani del Senato della Repubblica che periodicamente ci

Senatore Marcenaro, innanzitutto la Presidenza le formula i migliori auguri di buon lavoro per l'inizio della sua attività istituzionale, che abbiamo appreso avrà luogo nella giornata di oggi.

dell'istituzione di un premio annuale del Senato sui diritti umani. Ritengo l'iniziativa molto apprezzabile e confido sulla condivisione unanime dell'Assemblea su questo argomento.

si sarebbe potuto pensare che quel giorno segnasse l'inizio della sua applicazione, che coloro che avevano voltato la dichiarazione applicassero quei diritti nei rispettivi Paesi.

perché individuò il punto focale dal quale derivano la necessità e il convincimento di applicare i diritti umani, il riconoscimento della piena dignità e del valore assoluto dell'individuo. È un fatto assai significativo perché cioè avvenuto a metà del secolo scorso, un secolo nel quale ideologie che negavano la dignità dell'individuo, hanno originato le peggiori mostruosità compiute nei confronti di intere popolazioni, di intere categorie sociali, di milioni e milioni di persone che sono state uccise, private dei loro diritti e della loro libertà.

Molti Paesi che sono stati atroci dittature sono diventati democrazie; altri Paesi hanno conquistato la loro indipendenza spesso - ahimè, soltanto spesso e non sempre - garantendo questi diritti ai loro cittadini.

di tutti i Paesi che sottoscrissero quella dichiarazione impegnarsi ogni giorno per far progredire i diritti umani, a cominciare naturalmente dal proprio interno, ma promuovendoli a livello internazionale.

citare per esempio le gravi difficoltà che incontrano gli immigrati che vengono nel nostro Paese e magari ignorare fenomeni immensi come quelli che avvengono in Cina, dove - altro che le difficoltà che incontrano i nostri immigrati! - gli stessi cittadini di quel Paese sono ogni giorno privati in modo radicale della loro libertà. Le difficoltà sono anche di altro genere. I Governi naturalmente devono trattare con i Governi di tutti i Paesi e hanno il dovere di trattare anche con quelli dei Paesi che negano i diritti umani. In questo quadro i Parlamenti svolgono una funzione molto importante, perché non hanno questa relazione diretta con gli altri Paesi e, se ce l'hanno, ce l'hanno attraverso organismi interparlamentari nei quali è possibile dire quello che per un Governo diventa più difficile. In questo ambito il Gruppo del Popolo della Libertà nei pochi mesi di legislatura

finestra") contro le persecuzioni dei cristiani e la negazione della loro libertà; ricordiamo che la libertà religiosa è una delle principali libertà che vengono garantite dalla Dichiarazione universale.

nei confronti di quei rapporti economici che a volte rendono timidi gli organismi governativi nelle relazioni internazionali. Siamo convinti che il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dell'individuo sia anche una garanzia di progresso economico, una garanzia rispetto alle relazioni economiche e commerciali fra i Paesi. Il Gruppo del Popolo della Libertà continuerà con un impegno giornaliero, con la presentazione di documenti e con un'attenzione continua al riconoscimento dei diritti umani in Italia e soprattutto nei tanti Paesi del mondo in cui essi sono brutalmente negati.

Signora Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto vorrei ringraziare i relatori Saia e Pichetto Fratin e il relatore di minoranza Rossi Nicola, nonché tutti gli intervenuti in questo dibattito che è stato breve ma denso di contenuti. Si è parlato principalmente della crisi mondiale e poi delle misure che sono state adottate nel nostro Paese per farvi fronte. Certo, la crisi è di dimensioni inconsuete, per certi aspetti ignota, e quindi spaventa, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura perché fino adesso l'Italia, l'Europa e gli altri Paesi del mondo si sono mossi con razionalità, secondo un percorso a volte, nei casi principali, concertato a livello mondiale, mostrando che esiste una *governance* complessiva, anche se, certo, forse a livello europeo un passo in più sarebbe stato auspicabile. Si è riusciti comunque ad affrontare gradualmente la crisi, secondo le diverse contingenze che man mano si presentavano, a cominciare dalla crisi del credito. Certo, la crisi è anche l'occasione per ripensare fino in fondo le nostre strutture economiche e il nostro modo di essere. In qualche modo occorre rimettersi in gioco, occorre valutare ciò che è bene e ciò che è male nel nostro sistema, senza però rinunciare al nostro livello di civiltà, considerando, per esempio, che molte misure che sono state adottate, che magari verranno adottate e che, per certi aspetti, si avvicinano ad un meccanismo di statalismo derivante solo dalle contingenze immediate, comunque non possono farci abbandonare la linea Grazie, È stato osservato da parte di alcuni che le manovre operate dal Governo avrebbero in qualche modo una caratteristica prociclica, cioè volta ad esasperare ciò che sta accadendo. In realtà, non è così. Quelle Quelle adottate nel nostro Paese non sono manovre procicliche perché in qualche modo pongono al vertice, al centro di tutto la necessità di impostare una finanza pubblica rigorosa nella quale la diminuzione della spesa pubblica consenta, una volta superato il momento di crisi, di avviare quel processo di sviluppo che è pur sempre indispensabile per modificare la struttura della finanza pubblica e, quindi, dell'economia italiana. Altrimenti, se noi adottassimo altri tipi di misure, diciamo francamente anche un po' meno ortodosse rispetto a quelle che stanno assumendo i Governi europei e il Governo italiano, si correrebbe il serio rischio di un avvitamento tra la spesa, il deficit, ancora una volta la spesa e ancora una volta l'aumento della pressione fiscale. In sostanza, si darebbe, nel senso vero e proprio, avvio ad un meccanismo di recessione che ci porterebbe lontano e questo, sì, sarebbe difficilmente rimediabile. la crisi finanziaria rischia di innescare una crisi di economia reale, ma tale crisi di economia reale può essere contrastata con una serie di disposizioni e norme che man mano vengono adottate. adottate. Ripercorrendo molto rapidamente ciò che è stato fatto dal Governo italiano, non si possono dimenticare i due decreti sulle banche, che sicuramente non hanno la funzione di sostenere il settore bancario in sé, perché questo poco avrebbe senso,

qualche modo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, di creare un incremento di domanda e di rassicurare ancora di più i mercati e gli operatori economici, per esempio, le piccole imprese, con il sistema dei confidi.

aumentare la spesa o la spesa fiscale per almeno un punto di PIL in modo da dare ossigeno all'economia del Paese. Questo è un tema molto rischioso, anche perché in realtà

mentre da una parte ha dimostrato la necessità di svolgere un'azione concertata a livello europeo (cosa della quale peraltro si sente un certo bisogno), dall'altra ha detto che le singole economie devono provvedere, sempre però nell'ambito dei Patti di stabilità relativi a ciascun Paese.

Come Italia, dobbiamo attingere al debito pubblico, tanto è vero che per il prossimo anno abbiamo in bilancio 82 miliardi di euro come servizio del debito. È chiaro che, se andassimo ad un meccanismo di spesa non non controllata, di spesa crescente, e se i mercati vedessero che l'Italia non è in grado di tener fermo il timone della spesa, il rischio che il servizio del debito (cioè il costo del debito) aumenti, sarebbe molto alto. Ricordiamoci che già oggi subiamo un differenziale dei tassi rispetto al *bund* tedesco nell'ordine di 130-140 punti base. Il che vuol dire che paghiamo

Grazie. meccanismo di spesa sarebbe inteso semplicemente come fatto che adesso si spende di più. E un domani saremmo costretti ad inseguire con le tasse questo aumento di spesa, sostanzialmente sottraendo, dal circuito dell'economia e della produzione, delle risorse destinate a pagare il servizio del debito. Di conseguenza ci sarebbe un ulteriore incremento del costo del debito. Ogni manovra fatta sostanzialmente in deficit non riuscirebbe a ripagarsi con un aumento dello sviluppo dell'economia, ma si ripagherebbe con un ulteriore costo del debito, con il rischio di con il rischio di un avvitamento che non ci possiamo assolutamente permettere. In queste circostanze di difficoltà si pone qualche domanda di carattere generale. Per esempio, se sia il caso di adottare politiche più Il senatore Nicola Rossi, nella sua replica, ci ha invitato a fare attenzione, sottolineando il fatto che, camminando con lo sguardo a terra, si rischia di non guardare l'orizzonte e di non andare da nessuna parte.

considerazioni di prudenza, che capisco essere meno invitanti, anche dal punto di vista intellettuale, forse sono necessarie in circostanze difficili come queste, tenendo presente che le economie italiana ed europee si muovono comunque entro vincoli e condizioni molto strette che sarebbe difficile riuscire ad evitare. Il motivo che ho illustrato prima, con principale riferimento alla questione del costo del debito, e il rischio che in un sistema così volatile dei tassi e di mercati bancari possano esservi delle esplosioni dei tassi inducono a a mantenere una stretta linea di prudenza. Certo, altro è il discorso che, mentre cerchiamo di risolvere il problema della crisi attuale, non sia il caso invece di guardare in prospettiva alle riforme di struttura che potrebbero un domani, una volta finita la crisi, consentire a

in realtà la crisi, l'aumento della spesa pubblica, l'aumento delle tasse, le misure sbagliate che si possono prendere rischierebbero di pregiudicare di più le ragioni degli strati migliori o di quelli più svantaggiati della popolazione? assolutamente convinto che una politica scarsamente rigorosa rischierebbe di rovinare più i poveri che non i ricchi.

la spesa pubblica in aumento o in *deficit* non sia la via giusta e che la via del rigore economico sia quella migliore per salvaguardare questo tipo di interessi. Sono state avanzate poi alcune critiche circa lo strumentario adottato dal Governo. In sostanza ho sentito come aleggiare un rimpianto dei bei tempi andati, quando nella finanziaria *omnibus* si compendiavano tutti i desideri, tutte le aspirazioni; una sorta di

ed è stato detto in quest'Aula - qualche vena, non dico di rigore, ma di serietà nell'approccio ai conti pubblici è stato dimostrato dal Parlamento. Per fortuna è finita l'epoca nella quale si pensava di risolvere qualche problema semplicemente con un emendamento o con una modifica alla legge finanziaria. tempo sembra essere concluso, speriamo definitivamente. Sta di fatto che il meccanismo della finanziaria, come siamo abituati a considerarla, non esiste più, perché adesso la finanziaria è esclusivamente un un luogo nel quale si fissano i saldi e gli obiettivi complessivi di politica economica, lasciando ad altri interventi legislativi la definizione delle misure di dettaglio o settoriali. Questo ha consentito di rendere il meccanismo di finanza pubblica italiana molto più, se vogliamo, efficiente, stabile ed un vero punto di riferimento per tutta la legislazione

il decreto-legge anticrisi, il n. 185 della settimana scorsa, non copre la maggiore spesa in deficit ma la copre all'interno delle risorse previste in finanziaria, manifestando ancora una volta l'intenzione del Governo di intervenire, certamente sì, ma nei limiti delle risorse disponibili, senza eccedere la spesa pubblica e quindi senza creare quel rischio che sarebbe potuto derivare se avessimo assunto un diverso approccio. Questa è la nostra linea di politica economica: interventi sì, ma, ai sensi

quando si crearono le cause dell'attuale malessere, cioè spendere a debito, spendere condannando le generazioni future a pagare i debiti fatti. la finanziaria è il centro di riferimento di un sistema normativo stellare ed essa, seppur non sia più quella di prima, resta sempre l'atto più importante sotto il profilo della politica economica.

sarei più propenso a considerarli come una riconsiderazione dinamica della spesa, perché non sempre si tratta di tagli, a volte si tratta di aggiustamenti per particolari categorie di spesa. Quindi, ci sono state lamentele per le riduzioni di spesa sono state avanzate richieste di aumento di spesa per questo o quel settore. Mi rendo conto che molti settori manifestano esigenze di incremento di spesa, molti settori sono sensibili, però dobbiamo farci carico di una questione di carattere generale: non si può

Non esiste la possibilità di un *free ride* nella riduzione della spesa pubblica: tutti, in un modo o nell'altro, devono parteciparvi. Certo, vi è stata una lamentela circa il fatto che si sarebbero prodotti, soprattutto con il decreto-legge n. 112, tagli di natura orizzontale.

adottato in base al principio secondo il quale tosando la spesa si sarebbe affamata la bestia e quindi si sarebbero indotti i decisori pubblici a privilegiare la spesa necessaria e a sacrificare la spesa cattiva. Questo è il principio che sostanzialmente sta alla base del ragionamento di qualunque buon padre di famiglia: se diminuisco i miei redditi riduco le spese superflue e lascio la spesa laddove In realtà, l'operatore pubblico non opera come un padre di famiglia, lo abbiamo scoperto negli anni in cui abbiamo attuato questo tipo di esercizio: si è realizzata una sorta di legge di Gresham della spesa pubblica per cui la spesa cattiva scaccia la spesa buona; sono rimaste le spese cattive e sono state ridotte le spese buone, le spese buone, nella speranza, o nella convinzione, che prima o poi sarebbe intervenuto lo Stato a finanziare la spesa buona, i servizi indispensabili per la cittadinanza. Ciò ovviamente non funziona e non è condivisibile. Quest'anno non abbiamo più un sistema di tagli orizzontali della spesa ma, grazie all'articolo 60 del

molto importante, che non è più quello di andare al Tesoro a chiedere soldi ma di ragionare su come utilizzare razionalmente le risorse affidate al loro Dicastero, concentrandole sulla spesa buona e cercando di tagliare la spesa cattiva. Ovviamente, questo tipo di ragionamento non vale solo per i Ministri ma anche

nel testo approvato in Commissione al Senato è stato, per così dire, elasticizzato per consentire al limite più alto possibile l'utilizzo delle risorse disponibili per investimenti. E tutti sappiamo che in questa fase gli investimenti degli enti locali hanno anche una funzione anticiclica che va assolutamente assicurata.

di tagli orizzontali non avremmo neanche fatto interventi come quelli, ad esempio, sulla scuola. L'intervento di riduzione del costo della scuola,

che nella *spending* *review* dell'anno scorso e di quest'anno invitava il Governo a ridurre il numero dei plessi scolastici e a valutare la congruità del numero degli insegnanti di sostegno ed il rapporto tra insegnanti e alunni nelle nostre scuole.

di una volta, e sulla necessità, condivisa in molti interventi, di ristrutturare la legge di contabilità, facendo della legge di bilancio il perno fondamentale della politica finanziaria del Paese. La legge

triennalizzando il bilancio e quindi dando una prospettiva di stabilità ai nostri conti, facendo sì che il meccanismo della costruzione del bilancio per programmi e missioni assuma una base normativa, oltre che fattuale,

Mi domando poi se non sia il caso di passare ad un sistema di bilancio di cassa, più realistico rispetto al bilancio di competenza che attualmente abbiamo, che sostanzialmente lega le postazioni di bilancio più alle intenzioni che alla realtà. È ovvio che deve esservi un maggiore coordinamento tra i vari soggetti

estratti a consuntivo principalmente sulla base di elaborazioni dell'ISTAT, senza che il Parlamento, che è il luogo della sovranità, partecipi alla definizione dei dati stessi.

nelle ricette, nelle soluzioni e negli obiettivi. Con questo spirito ringrazio l'Aula del Senato, auspicando una rapida approvazione dei disegni di legge al nostro

Le modifiche apportate in Commissione, com'è evidente, sono del tutto marginali, se si eccettua la norma di integrazione del finanziamento del sistema scolastico:

che dovrebbero, a nostro modo di vedere, essere contenute in questi provvedimenti, ma segnaleremo anche problemi puntuali, urgenti e non rinviabili. Lo abbiamo già fatto in Commissione molto spesso il relatore e il Governo hanno riconosciuto la fondatezza delle nostre argomentazioni, ma opponendo o un rifiuto non motivato oppure rinviando le questioni ad altri provvedimenti legislativi. proposito introduco una riflessione più generale per poi formulare una richiesta sull'ordine dei lavori. Il Governo si vanta - lo ha detto poco fa il sottosegretario Vegas - di aver svuotato o comunque ridotto l'ambito di operatività dello strumento della legge di di bilancio, di aver superato il sistema delle finanziarie *omnibus*. In realtà è intervenuto semplicemente un frazionamento degli strumenti, tant'è vero che è dall'inizio della legislatura ci stiamo

una discussione ampia e libera da condizionamenti temporali. Più volte, signora Presidente, abbiamo denunziato lo svilimento dell'attività parlamentare in generale: molte volte non c'è ascolto, si oppongono pareri contrari senza nessuna motivazione, la maggioranza è ridotta a ratificare

i provvedimenti tra maggioranza e Governo in modo tale che, appunto, si sancisca in via definitiva che il Parlamento può dire solo sì o solo no. Ecco, questo è il quadro, questa è la situazione. All'interno di tale quadro e a fronte di una manovra complessivamente intesa, con tutti gli strumenti che richiamavo, assolutamente corposa in termini quantitativi ma anche per contenuti delle norme di legge approvate, a fronte dei problemi che il Paese si trova ad affrontare, della grave crisi (la più grave dal dopoguerra), con evoluzioni continue che a volte rendono evidente che gli strumenti, le decisioni e i provvedimenti adottati sono superati

nell'esprimere i pareri sugli emendamenti svolgano le loro motivazioni - favorevoli o contrarie - con prese di posizioni precise, chiare, esaustive. C'è tempo, c'è tutta la settimana per fare in modo che si faccia un lavoro serio - noi non vogliamo fare alcun ostruzionismo - e che ci si predisponga non soltanto a dire dei no. In questi

che il decreto-legge n. 112 arrivi al Senato della Repubblica in tempo utile e in condizioni tali da consentire lo svolgimento di una discussione, anche in questo caso, approfondita e priva di condizionamenti. Mi auguro che questo richiamo e queste invocazioni vengano ascoltate dal Governo, dai relatori e dalla maggioranza. *(Applausi

La Presidenza, da parte sua, farà di tutto per assicurare un confronto certamente franco, ma sereno e costruttivo. Sull'ultimo punto riferirò al presidente Schifani.

Signora Presidente, naturalmente non entro nel merito della questione posta dal senatore Astore, perché è assolutamente condivisibile che si discuta un problema importante come quello da lui posto, ma voglio precisare in che termini sta la questione.

perché già negli anni precedenti non soltanto era presente in quest'Aula, già allora autorevole esponente della maggioranza, oggi opposizione, ma è stato altresì relatore della finanziaria. Ricordo a lui e a quanti erano presenti che già a quel tempo io mi esposi più volte a chiedere che il relatore facesse, nell'espressione del parere, un riferimento agli elementi sostanziali presenti nella richiesta emendativa.

In questa fase della discussione, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 129 del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli e quindi il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere. Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge finanziaria.

parere di nulla osta». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3002, 2.3003, 2.3004, 3.Tab.A.28, 2.3, 2.6, 2.27, 2.28, 2.49, 2.112, 2.137, 2.182, 2.183, 2.188, 2.189, 2.227 e 2.546. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

In particolare questi emendamenti riguardano la destinazione di una quota, pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base di dichiarazioni annuali, in parte a scopi di interesse sociale e culturale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopo di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Tali quote sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali e alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo. la detrazione dell'ICI per le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale,

che operano nell'ambito delle politiche migratorie, con particolare riguardo alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo. Inoltre, è prevista la stabilizzazione della misura a decorrere dal prossimo anno finanziario 2009 (con le dichiarazioni dei redditi relativi al 2008), al fine di il *welfare* non come un capitolo di spesa, ma piuttosto come una leva dello sviluppo, uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà attiva dei cittadini, sottraendo il flusso del 5 per mille delle leggi annuali di bilancio (rimasta finora affidata alle singole leggi finanziarie: commi 337 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266

a favore dei Paesi in via di sviluppo ed un accantonamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio della finanziaria, finalizzato a ripristinare le risorse per il «Programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», risorse ridotte nel bilancio 2009 rispetto a quanto previsto dall'assestamento di bilancio del 2008. L'approvazione di tale emendamento consentirebbe di ricostituire una notevole parte delle risorse tagliate ai capitoli di spesa che destinano risorse agli italiani all'estero e troverebbe copertura nella Tabella C, ossia nelle voci di spesa relative agli stati di previsione dei vari ministeri, con l'esclusione di alcune poste socialmente sensibili il ripristino dei tagli effettuati dal Governo per il «Programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali». di soggiorno legale necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale è stato introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008 per evitare che cittadini stranieri immigrati in Italia sulla base della semplice iscrizione anagrafica possano usufruire della prestazione assistenziale. Con questo emendamento si intende garantire, nel rispetto dei requisiti anagrafici e reddituali vigenti, l'assegno sociale ai cittadini italiani emigrati i quali rientrano definitivamente in Italia (l'assegno è subordinato alla residenza e non è esportabile o erogabile all'estero) e possono far valere almeno dieci anni di residenza cumulativi nel territorio nazionale in qualunque periodo della loro La copertura dell'emendamento è calcolata fino a un importo di 25 milioni di euro; secondo le quantificazioni un aumento del 10 per cento

la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale, ma anche in sede civile, tributaria e amministrativa. La seconda è che la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente, oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine, cui vanno assicurati mezzi indispensabili per il loro operato, un sistema giudiziario efficiente per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia. Invece, dobbiamo osservare che in questo disegno di legge di bilancio sono previste riduzioni molto pesanti e significative agli stanziamenti del Ministero della giustizia, che rappresentano soltanto l'1,4 per cento delle risorse totali del bilancio dello Stato, con una riduzione del 4,1 per cento rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, si registrano complessivamente riduzioni di stanziamenti di circa 32,5 milioni di euro, con decremento del 3,6 per cento rispetto alle previsioni della legge di assestamento. Tutte queste riduzioni interessano la missione giustizia rispetto al precedente esercizio finanziario e, in particolare, ammontano a 341 milioni di euro. Riduzione significativa e suscettibile di determinare un forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, quando non addirittura una sua paralisi tale da generare una situazione ulteriormente grave rispetto a quella attuale che è sotto gli occhi di tutti.

e parallelamente si registra il taglio dei cosiddetti consumi intermedi, cioè delle spese per l'acquisto di beni e servizi per il settore della giustizia civile e penale. Inoltre, si assiste ad una forte riduzione delle risorse destinate agli investimenti nell'ambito del medesimo programma, senza che vi siano stanziamenti sufficienti per la realizzazione del processo telematico, addirittura con una contraddizione con quanto afferma il Governo, in particolare il Ministro della giustizia, ripetutamente in pubblico. - riduzione dello stanziamento per il processo telematico, che viene qualificato invece come obiettivo prioritario, idoneo a determinare una significativa accelerazione dei tempi dei processi. La concretezza di questa manovra finanziaria ci dice che la maggioranza e il Governo si stanno muovendo in senso nettamente contrario. Per quanto concerne le ulteriori riduzioni al programma di giustizia minorile e all'edilizia giudiziaria penitenziaria e minorile interverranno altri colleghi in maniera specifica. Inoltre, si osserva un dimezzamento dello stanziamento per il funzionamento della scuola superiore della magistratura. Queste riduzioni vanno ad aggiungersi ai tagli che sono stati disposti con il decreto-legge n. 112 del 2008,convertito con la legge n. 133 del 2008: in esso era stato già disposto un taglio per il triennio che ammonta a circa il 40 per cento delle risorse destinate al Ministero della giustizia. quindi di proclamazioni sulla priorità dei comparti sicurezza e giustizia assistiamo invece a fortissimi decrementi, che renderanno questa macchina giudiziaria ancora più ingolfata e quindi incapace di rendere giustizia sostanziale e vera ai cittadini.

che viene ad incidere anche sulla giustizia minorile, comporta una fortissima compressione proprio di quei diritti umani di cui oggi abbiamo parlato nella celebrazione dell'anniversario della Dichiarazione fondamentale dei diritti umani. Sarà impossibile realizzare, nell'interesse delle madri detenute e quindi dei minori che sono detenuti involontariamente insieme alle madri, programmi che consentano effettivamente di attribuire condizioni di vita adeguate a un Paese civile. Sotto questo aspetto, sia per l'edilizia penitenziaria che riguarda le carceri minorili, sia per la possibilità di avere appoggi esterni attraverso case famiglia, sia per la possibilità di assicurare condizioni di vita adeguate ai minori, ritengo che questi tagli siano particolarmente pericolosi

e successivamente la triste vicenda Alitalia, dopo aver sottratto ingenti e preziose risorse in conto capitale già destinate a opere pubbliche e infrastrutture prevalentemente localizzate al Sud,

e questo alla faccia delle misure anticicliche paventate per contrastare l'imminente crisi economica, i cui effetti purtroppo devastanti cominciano pesantemente

illustrare solo alcuni emendamenti: altri colleghi dopo di me interverranno sulle risorse che sono state sottratte alle principali infrastrutture. Mi limito volutamente

la necessità di ripristinare le risorse che non sono state coperte per quest'anno, ma che in maniera particolare pregiudicano l'esercizio dei servizi di cabotaggio rivolti alle isole minori per i prossimi anni. Vogliamo sottolineare questi emendamenti perché siamo consapevoli che la situazione della Tirrenia non è la situazione dell'Alitalia; ma se il Governo continua nei suoi propositi, può davvero diventare un nuovo caso Alitalia. Vogliamo che il Governo riparta dal piano industriale presentato dalla compagnia Tirrenia, che - ricordo - prevedeva come obiettivo un processo di privatizzazione della compagnia, un risparmio

tutto questo nella completa assenza del Ministero del lavoro. Soprattutto il Governo deve fare chiarezza su cosa impone davvero l'Unione europea, per non prendere

rotte significative di collegamento dal continente alle isole minori vengano tagliate nel prossimo esercizio finanziario e soprattutto - come ci è stato detto dall'amministratore delegato Pecorini che questo comporti riflessi negativi per 400-500 posti di lavoro. Si tratta di un provvedimento molto contenuto, nell'ordine di 50-70 milioni di euro, che sicuramente avrebbe diversi benefici ed effetti.

Colleghi, per cortesia, vi invito a prendere posto, siamo in votazione, diventa difficile controllare anche per i colleghi senatori Segretari. **Il

Dichiaro aperta la votazione.

l'incongruenza della Tabella 3 in riferimento alla riduzione di risorse per il commercio internazionale, per il sostegno e la promozione del *made in Italy* e per la ricerca e l'innovazione tecnologica, oltre ad una riduzione di 271 milioni di euro per la competitività e lo sviluppo delle imprese. Con gli ordini del giorno intende impegnare il Governo ad agire perché quelle risorse vengano riallocate per missioni ed obiettivi che ci paiono particolarmente importanti soprattutto in questa fase.

Dichiaro aperta la votazione.

e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011", si rileva che gli stanziamenti del Ministero della giustizia, che rappresentano peraltro solo l'1,4 per cento delle risorse totali del bilancio dello Stato, registrano inopinatamente una forte riduzione rispetto all'esercizio precedente, che aveva già subito delle riduzioni. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2009 le risorse complessivamente stanziate per l'attuazione del programma relativo all'amministrazione penitenziaria sono decisamente insufficienti al perseguimento degli obiettivi scritti nel medesimo programma. Sono fortemente ridotti gli stanziamenti relativi al funzionamento dei servizi istituzionali e, tra gli altri, quello relativo ai servizi sanitari penitenziari e comunque del trattamento per l'intero processo detentivo. Credo che su questo punto la maggioranza dovrebbe porre la massima attenzione, perché non si tratta di andare incontro alle esigenze dei detenuti, ritenuti da molti degni di repressione Le risorse destinate esclusivamente alla tutela dei detenuti, che sono fortemente ridotte, non sono un privilegio da concedere alla massa dei detenuti (la definisco in questo modo, perché via via sta crescendo il numero dei detenuti).

per cui aumentando la repressione, aumenta la popolazione carceraria, e non è un fatto che riguarda solo i detenuti. Considerato, come più volte è stato indicato, che il Consiglio d'Europa ha ben evidenziato ben evidenziato che attraverso la pena detentiva si perseguono obiettivi di reinserimento sociale, aspetto che definirei di natura ideale o di valori condivisi a livello europeo, vi è un aspetto ancora

la pratica della gestione corretta e civile di questa popolazione carceraria, non facciamo un danno solo ai detenuti: c'è tutta la popolazione del corpo di polizia, degli educatori e di tutto il personale che lavora all'interno delle carceri che con questo sistema vedrà messe

Signora Presidente, volevo specificare che alla tabella 7, attraverso un emendamento presentato in Commissione, è stato introdotto il punto 1.14; di nuova

Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, avverto che con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno determinati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali. L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata preclusiva della discussione e della votazione di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati. Gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili. La valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame risulterà contabilmente nella Nota di variazioni

vorrei ricordare che ieri sera in quest'Aula i relatori, presentando le proprie valutazioni sulla discussione intorno alla manovra finanziaria, l'hanno giudicato, estremamente soddisfacente, perché disegnava il profilo di un'analisi condivisa della situazione economica del Paese. Credo che possiamo affermare che, se l'analisi è condivisa, certamente non sono condivise le soluzioni proposte per affrontare la crisi economica in cui versa il nostro Paese.

il CENSIS - capacità di adattamento reale ed incisiva capacità di innovazione. Condividiamo questa analisi ed è partendo da riflessioni coerenti con essa, e non solo con essa, che abbiamo proposto di affrontare la crisi con una manovra espansiva, dedicando un punto di PIL ad alcune importanti azioni di protezione sociale e di sostegno alla ripresa che giudichiamo indispensabili. In particolare, le misure proposte con l'emendamento 1.0.2 destinano oltre la metà di questo punto di PIL, di PIL, quindi un investimento importante, a migliorare la capacità reddituale delle persone e delle famiglie, diminuendo la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed aumentando le detrazioni fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti ed autonome, nonché di quelle occupate con contratti parasubordinati.

3,5-5 miliardi) viene destinato dalle nostre proposte all'alleggerimento della pressione fiscale sui redditi da lavoro e all'incremento della produttività attraverso la detassazione del salario derivante dalla contrattazione aziendale e, in generale, da quella di secondo livello. Ci riferiamo, quindi, ad un complesso di interventi di sostegno del reddito personale e, conseguentemente, del reddito familiare, con un valore strutturale, cioè con effetti permanenti sul reddito disponibile, e con un miglioramento dell'equità del sistema impositivo. Dunque, l'attenzione alla consistenza del reddito, alla condizione materiale della vita delle persone e delle famiglie ed alla conseguente - si badi, lo voglio sottolineare, conseguente a queste misure, non vagheggiata - possibilità di offrire uno stimolo alla ripresa dei consumi consumi è al centro della nostra proposta. Le ragioni che la motivano stanno nei numeri che nel corso dell'anno hanno delineato la situazione reddituale della maggioranza degli italiani. Sempre il CENSIS conferma che l'impoverimento relativo, cioè l'impossibilità di adeguare il proprio reddito all'aumento dei prezzi, riguarda ormai l'84,7 per cento della popolazione attiva. Il dato interessa in via assolutamente prevalente, cioè in misura superiore all'87 per cento, i redditi medio-bassi. La difficoltà di incrementare i propri redditi da lavoro correla in maniera diretta con la capacità di mantenere gli stessi livelli di tenore di vita di tre anni fa. Entrambi i dati, infatti, riguardano il 94,4 per cento degli occupati. Questo nonostante le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Il quadro che si prospetta per il 2009, secondo un recente studio di Confindustria, prevede che il consumo delle famiglie italiane rispetto all'anno precedente si ridurrà ulteriormente dall'attuale meno 0,2 per cento (dato del 2008)

14 milioni di lavoratori guadagnano meno di 1.300 euro netti al mese; di questi, 7,3 milioni ne guadagnano meno di 1.000. Questo consolida una situazione rispetto alla capacità di spesa delle famiglie che vede

che non riesce a riscaldare adeguatamente il proprio alloggio, il 4 per cento che non ha risorse sufficienti per le spese alimentari, oltre il 10 per cento che non riesce a garantirsi le spese mediche non coperte dal sistema sanitario, oltre il 16 per cento risorse sufficienti per l'abbigliamento. Le cause di questa situazione sono molteplici. Innanzitutto il differenziale rilevantissimo tra l'indice ISTAT rilevato e l'indice ISTAT programmato, sul quale poi si vanno a stabilizzare i rinnovi dei contratti di lavoro.

derivanti da contrattazione integrativa o comunque da premi legati alla produttività, proponiamo un incremento delle detrazioni fino al 23 per cento. Da ultimo vorrei richiamare quanto previsto all'emendamento 1.0.5 in termini di

Proporre l'incremento delle detrazioni a favore delle donne occupate, quale che sia la loro forma di occupazione, quindi a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, non solo mira a ridurre il differenziale reddituale tra uomini e donne, ma, rapportandosi al numero dei figli, si propone di riconoscere il carico di cura che le donne sostengono alla maternità e di veicolare il sostegno al reddito familiare per il tramite delle lavoratrici, con ciò garantendo che la valorizzazione del reddito familiare non si trasformi in disincentivo

I senatori che vogliono seguire la discussione la seguano, altrimenti escano, perché la Presidenza non ha capito niente. Vorrei sapere quanti in quest'Aula hanno potuto seguire l'illustrazione della senatrice Ghedini. La Presidenza invece vuole seguire e far seguire i senatori che vogliono svolgere il proprio ruolo.

con qualche pretesa di completezza e di precisione, signori del Governo, collega relatore e colleghi della maggioranza, alla domanda che ogni opposizione seria, che aspiri credibilmente a conquistare i consensi della maggioranza del popolo, deve rivolgere a se stessa e deve sempre accettare che le venga rivolta dall'esterno. La domanda è la più banale: «Ma voi, al posto loro, cosa fareste»? Questa risposta l'emendamento la dà, riconoscendosi in partenza un limite: gli emendamenti alla legge finanziaria, per essere ammessi, debbono essere compensati dentro i saldi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa risoluzione.

Se fossimo al Governo avremmo presentato una Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, nella quale avremmo programmato scientemente un peggioramento di un punto nel rapporto indebitamento/PIL nell'anno 2009, prevedendo l'immediata adozione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di interventi legislativi ed amministrativi capaci di ridurre la spesa corrente primaria per entità crescenti nel 2010, 2011 e 2012 fino al pareggio di bilancio, così come previsto dal Patto di stabilità e di crescita presentato e sottoscritto in Europa dal Governo Prodi e, dico subito, meritoriamente per allora accettato anche dal Governo Berlusconi. Dunque, man mano che sentirete avanzare le nostre precise proposte, le dovrete pensare collocate in questa cornice di politica fiscale e di bilancio. Una politica di bilancio a cui noi nel 2009 daremmo una intonazione responsabilmente espansiva mentre voi, il Governo e la maggioranza, pretendete di mantenerla come una politica di bilancio duramente restrittiva. Detto questo, perché senza questa premessa la nostra proposta non può essere compresa nella sua effettiva sostanza, veniamo all'illustrazione dell'emendamento in esame. le chiedo di avere un po' di comprensione per la vastità e la completezza della proposta che in questa sede avanziamo. Con l'articolo 1-*bis* disponiamo un aumento della detrazione IRPEF sui redditi da lavoro dipendente. Di tutte le misure che proponiamo, questa è certamente la più onerosa dal punto di vista dei suoi effetti sul bilancio. È volta ad aiutare le famiglie (percettori di reddito) con reddito medio-basso. Trasforma - questo è un punto molto importante della nostra proposta - la detrazione in assegno nel caso di reddito incapiente. È una misura strutturale di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro medio-bassi. È una misura, quindi, di carattere permanente e per questo, a nostro avviso, può davvero accompagnare, e in una misura non rilevantissima, determinare un aumento dei consumi delle famiglie.

Per basso che sia il reddito di una persona, colleghi della maggioranza e del Governo, se quella persona pensa che il domani sarà peggiore dell'oggi e riceve dieci euro in più,

ma di risparmiarla per quando la situazione diventerà peggiore. Non è una scelta irrazionale. Al contrario! È una scelta perfettamente razionale che una persona, in una situazione di prevedibile peggioramento della sua condizione, fa quando riceve un piccolo alleviamento alle sue condizioni di difficoltà. Per quello che riguarda l'articolo 1-*ter*, passiamo da una proposta di riduzione della pressione fiscale di tipo generalizzato - cioè che ha di fronte una platea amplissima di contribuenti, come nel caso che ho appena illustrato ad una proposta quantitativamente e qualitativamente più selezionata. In buona sostanza, proponiamo di detassare in modo significativo la quota di salario da contrattazione di secondo livello. Certamente si tratta anche in questo caso di una proposta volta ad affrontare la tragedia che chiamiamo questione salariale, cioè salari che crescono troppo poco oppure che non sono cresciuti affatto, questa proposta ha ambizioni di riforma strutturale. È un intervento che vuole avere un effetto anche nell'immediato, anche nei primi mesi del 2009, ma ha ambizioni di tipo strutturale. Ora, voi sapete, colleghi, che è in corso da molto tempo, ed è entrata su qualcosa di molto simile ad un binario morto, la trattativa per la riforma del modello contrattuale.

Da allora utilizziamo un modello contrattuale che non è efficace, né come strumento di politica redistributiva, né come strumento per affrontare la tragedia della

per la riforma del modello contrattuale e poi sviluppate una trattativa a livello aziendale, territoriale, di distretto o di filiera produttiva, io Stato Stato ridurrò la pressione fiscale su quella quota di salario che avrete inserito nella contrattazione di secondo livello», in modo tale da esaltare il ruolo della contrattazione di secondo livello

il primo passo (non esaustivo, naturalmente) per la costruzione in Italia di un sistema universale di ammortizzatori sociali, cioè di un sistema di sostegno del reddito e di promozione e di promozione e di aiuto del lavoratore nella sua ricerca di lavoro (quando lo perde o quando non ce l'ha), che in Italia presenta caratteristiche arcaiche. La cassa integrazione guadagni, così come è stata pensata molti decenni orsono, è totalmente inefficace nel rispondere all'esigenza di protezione dei lavoratori più deboli

colleghi della maggioranza, quando un sistema universale di ammortizzatori sociali? Se non adesso, quando? Nel 2009 voi sarete costretti - lo state già facendo, anche su sollecitazione nostra e delle parti sociali, a concedere centinaia e centinaia di milioni di euro di risorse per la cassa di integrazione in deroga, come si dice in gergo tecnico.

dopo aver speso un miliardo di euro per cassa integrazione in deroga, ritrovandoci alla fine esattamente il sistema di ammortizzatori sociali sperequato e profondamente inefficace che abbiamo adesso e che manteniamo da

basta ai contributi concessi sulla base della domanda, della raccomandazione, della sollecitazione, perché questo produce cattiva economia e cattiva politica. Proponiamo dunque una riduzione drastica del volume dei contributi a pioggia alle imprese, con una

Oggi il sistema delle imprese (tutte comprese, ma in particolare, come al solito, quelle piccole, piccolissime e medie) soffre di una crisi di liquidità. Il credito è difficile da trovare, non sempre le garanzie che vengono richieste ci sono. Questo problema si

dotate di formazione professionale e culturale adeguata che sono talmente deluse circa la possibilità di trovare impiego che non scendono nemmeno sul mercato del lavoro. Si parla, in termini di scienza economica, di livello della partecipazione alle forze di lavoro. vogliamo incentivare la partecipazione delle donne alle forze di lavoro, come sempre diciamo, perché così dispone il Trattato di Lisbona, bisogna fare Lisbona, bisogna fare in modo che la pressione fiscale sul reddito percepito e sul costo del lavoro di una donna per l'impresa sia inferiore a quella che, a lavoro e reddito equivalenti, deve essere sopportata da un lavoratore maschio e dall'impresa che impiega un lavoratore maschio. Si tratta di una proposta di portata straordinaria perché introduce una differenziazione che

valutazione di tutte le pubbliche amministrazioni, valutazione di ogni singolo aspetto e valutazione di ogni singolo dipendente o dirigente delle pubbliche amministrazioni. luogo, *benchmarking* o comparazione sistematica, fondata sulla valutazione precedente dei risultati e dei costi sopportati da ogni segmento della pubblica amministrazione, in maniera tale da rendere da rendere credibili obiettivi di risparmio e di riqualificazione fondati non su astratti disegni di ristrutturazione, ma sulla concretezza dei risultati raggiunti dalle parti migliori della pubblica amministrazione stessa. luogo, responsabilità ovvero obiettivi precisi di *performance* e di costo - e dunque di risparmio - ai quali associare, sulla base della verifica dei risultati, il premio oppure la penalizzazione.

Altrimenti i tagli orizzontali produrranno ciò che hanno sempre prodotto, vale a dire continueranno a penalizzare le amministrazioni migliori, che quello che bisognava fare per ristrutturare e riqualificare lo hanno già fatto, e continueranno a lasciare inalterate le possibilità di spreco delle amministrazioni peggiori. *(Applausi dai Gruppi PD e

gli emendamenti a mia prima firma presentati a questo articolo riguardano due temi molto strettamente collegati fra di loro che noi riteniamo di straordinaria importanza per lo sviluppo del Paese, anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.

Sappiamo che si tratta di temi ostici per questo Governo, che sono problemi verso i quali i Ministri competenti dimostrano scarsa o nessuna sensibilità, ma noi ci ostiniamo ugualmente a presentare le nostre proposte e i nostri emendamenti, perché siamo convinti che che proprio nell'occupazione femminile - lo richiamava poco fa il senatore Morando - risieda una straordinaria risorsa per la ripresa e la crescita economica e, vorrei aggiungere , civile del nostro Non posso e non voglio pensare che il Governo, nelle persone dei ministri Tremonti, Sacconi, Carfagna non stia monitorando il mercato del lavoro e non sappia che questa crisi economica finirà per pesare in gran parte sulle spalle e sulle vite delle donne, le quali - lo sappiamo tutti - svolgono i lavori più precari, sono quelle più esposte alla perdita del posto di lavoro, alla cassa integrazione, alla precarietà, alla povertà. E allora, qual è l'atteggiamento del Governo? Assecondare questo processo di impoverimento oppure sostenere le donne a rischio? E cosa pensa la ministra Carfagna? Non abbiamo sentito da lei, purtroppo, una sola parola di dissenso rispetto alla linea Tremonti-Sacconi. Le va bene tutto? Le va bene che questa legge finanziaria, come gli altri provvedimenti approvati finora, non preveda un solo euro destinato a portare avanti il piano per nuovi asili nido avviato dal Governo Prodi? Le va bene che si lasci cadere il Fondo di sostegno all'imprenditoria femminile, che non vi sia una sola proposta per sostenere politiche attive a favore dell'occupazione femminile, che non venga in alcun modo riconosciuto il lavoro di cura e che le donne continuino ad essere costrette a lasciare il posto di lavoro quando nasce il primo figlio? Le va bene che nel Sud l'occupazione femminile sia ormai al di sotto del 25 Altro che obiettivo di Lisbona al 60 per cento entro il 2010! Con i nostri emendamenti, signori del Governo, noi proponiamo di cominciare ad invertire la tendenza prevedendo alcune misure, alcune delle quali sono già state illustrate dai colleghi del mio Gruppo. Io ne voglio richiamare cinque. In primo luogo proponiamo una proroga e l'incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno. La seconda proposta riguarda la riqualificazione e il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

prevediamo detrazioni fiscali delle spese sostenute dalle famiglia per l'assistenza ai bambini e agli anziani ed infine quinta proposta, lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Sono misure che disegnano un welfare moderno, basato sulla persona, perché questo è ciò di cui abbiamo bisogno per valorizzare la risorsa femminile, per dare valore alle competenze, alle professionalità, alle abilità delle donne. È davvero un peccato, signor Sottosegretario, mandare sprecata questa risorsa. Noi non lo vogliamo e per questo insisteremo con le nostre proposte.

Ringrazio il Presidente e saluto il rappresentante del Governo, che ha già avuto modo in altre occasioni di ascoltarmi in merito all'emendamento che propongo, l'1.0.11, relativo al Patto di stabilità. Questo emendamento si pone come obiettivo quello di modificare il meccanismo del Patto di stabilità per i Comuni sopra i 5.000 abitanti. Non si tratta di un emendamento con fini ostruzionistici o di norme che gravano sui vincoli fissati dal Trattato di Maastricht. Anzi, tutt'altro! L'Unione monetaria pone due vincoli per l'insieme delle pubbliche amministrazioni: che il deficit non superi il 3 per cento del prodotto interno lordo e che come obiettivo arrivi al pareggio di bilancio, mentre per l'indebitamento l'obiettivo è che questo non superi il 60 per cento del PIL. In questi anni il Patto di stabilità applicato agli enti locali è stato fatto con meccanismi che si sono concentrati sul blocco della spesa e sul miglioramento dei saldi, con l'attenzione rivolta soprattutto al parametro del deficit. Meccanismi sicuramente validi per quella parte della pubblica amministrazione che non ha l'obbligo del pareggio di bilancio. Nella costruzione dell'emendamento abbiamo tenuto conto di due elementi fondamentali: il primo è che le norme contabili, a cui sono soggetti gli enti locali, non permettono di produrre deficit; infatti, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio. Il secondo è che gli stessi enti per la spesa in conto capitale possono far ricorso al credito e quindi con il loro comportamento contribuiscono all'incremento o al decremento dell'indebitamento della pubblica amministrazione. Il meccanismo del Patto di stabilità, che prende come parametri i valori relativi alla spesa e ai saldi degli anni precedenti, è un sistema perverso: penalizza eccessivamente gli enti virtuosi e di fatto non "morde" gli enti inefficienti e spreconi. Se consideriamo poi che negli anni scorsi sono state tolte le sanzioni per i Comuni che non avevano rispettato il Patto di stabilità, comprendiamo benissimo che vi è una vera e propria ingiustizia. Gli enti che hanno sempre rispettato le norme sono penalizzati, mentre quelli che non le hanno rispettate di fatto sono stati premiati. Il meccanismo del Patto di stabilità applicato agli enti locali in questi ultimi anni ha posto vincoli alla spesa corrente indipendentemente dalle entrate proprie. A partire dal 2007 ha previsto il miglioramento dei valori dei saldi di bilancio rispetto agli anni precedenti. L'insieme di queste norme ha prodotto nel corso degli anni le seguenti distorsioni: l'introduzione della finanza creativa anche per gli enti locali, al solo scopo di rispettare il Patto di stabilità; il ricorso a strumenti finanziari anomali come i derivati; le esternalizzazioni di molti servizi, soprattutto di quelli che avevano maggiori entrate proprie; un rallentamento dei pagamenti, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, allo scopo di centrare l'obiettivo del Patto di stabilità per cassa, con effetti negativi diretti sull'economia reale. L'attenzione dello Stato rivolta soprattutto al deficit e alla spesa corrente ha distolto l'attenzione dal valore del indebitamento degli enti locali, che dal 1998 al 2007 è passato dal 1,5 per cento al 3,5 per L'emendamento da noi proposto non vincola gli enti locali ai parametri del passato ma è un meccanismo dinamico che guarda avanti e che pone, come obiettivo primario, che i Comuni contribuiscano alla riduzione dell'indebitamento della pubblica amministrazione e che procedano verso una qualificazione della spesa, oltre che verso una maggiore responsabilità, in quanto considera più virtuosi e responsabili gli enti che hanno una maggiore autonomia finanziaria. È un È un meccanismo assolutamente diverso, saggio e meritocratico e, in questo senso, propone più equità, più giustizia, più responsabilità, più autonomia, un minor indebitamento della pubblica amministrazione e meno sprechi e inefficienze.

forza molto superiore rispetto a quella che non avrebbero avuto se fossero state iniziative isolate o corrispondenti solo a una volontà della maggioranza. la tematica complessiva degli emendamenti illustrati dal senatore Morando è condivisibile nello spirito; magari c'è qualche dettaglio non del tutto condivisibile ma questo è, per l'appunto, un dettaglio. La questione è prevalentemente di sede, nel più o meno condivisibile, ma se la scelta del Governo è stata quella di varare una finanziaria in cui si illustrano sostanzialmente solo i saldi per poi dedicare un altro provvedimento agli interventi di sostegno dell'economia,

ove vi siano - con il contenuto del provvedimento governativo. Quindi, sotto questo profilo, francamente l'invito che mi permetto di rivolgere ai presentatori è di ritirare gli emendamenti confluiti nell'1.0.1-*bis* per discuterli in quella sede, altrimenti allo stato il parere non può essere positivo per i motivi che mi sono permesso di illustrare.

principali problemi è quello di una produttività troppo scarsa rispetto ai nostri concorrenti. Faccio presente che così come è previsto il meccanismo, anche se anche se è molto sponsorizzato dalla parte sindacale, sostanzialmente consente che aumenti di reddito non siano tassati. Allora mi chiedo perché questo debba valere solo per i lavoratori e non anche per i pensionati o per altri tipi di soggetti. È un problema che io mi porrei.

Mi sento di acconsentire meno sull'articolo 1-*septies* perché, laddove si riducono i trasferimenti in conto capitale alle imprese, in certi casi questo può essere giustificato, ma in altri - per esempio per le imprese pubbliche - sarebbe contraddittorio.

di grande interesse. Ovviamente, siccome le lavoratrici, per essere congruamente incentivate, devono avere un vantaggio fiscale visibile, è evidente che si pone anche qui un problema di copertura Parte della copertura degli emendamenti dell'opposizione trae linfa dall'istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni. Mi permetto solo due rilievi di carattere generale, posto che lo strumento potrebbe anche funzionare, ma lo si vedrà solo *a posteriori*. del meccanismo di rinviare la decisione. Ora, mi rendo conto che talvolta le decisioni non si prendono e quindi trovare un meccanismo adeguato di rinvio può risolvere il problema, ma non vorrei che diventasse una sorta di clausola di stile, come quando si usava

canali e degli oggetti di riduzione della spesa pubblica: credo che la politica debba avere il coraggio di scegliere direttamente dove andare a toccare e tagliare, altrimenti, francamente, mi chiedo cosa stiamo a fare noi tutti qua

la questione del credito d'imposta per l'occupazione femminile nel Mezzogiorno. Il credito d'imposta sarebbe uno strumento di per sé molto utile, perché agisce immediatamente; il fatto di non averlo plafonato ha provocato sfondamenti di spesa non programmati e questo sicuramente non è condivisibile. Dunque il meccanismo del credito d'imposta in funzione di sviluppo di per sé sarebbe bello, perché esclude la discrezionalità amministrativa, ma praticamente fa correre il rischio di un eccesso Invece, qui e adesso, non dico in un futuro, ma nelle condizioni economiche in cui ci troviamo, condividere l'estensione dei congedi parentali francamente mi sembra fuori fuori rispetto alle necessità dei tempi. Posso condividere lo spirito della norma, ma non nel momento in cui in qualche modo dobbiamo andare a stringere la spesa in tutti i settori. L'ultima questione riguarda il Patto di stabilità interno, illustrata dal senatore Stradiotto. È chiaro che il meccanismo di definire premi e sanzioni e distinguere tra enti virtuosi ed enti meno virtuosi meno virtuosi è essenziale per superare il sistema che sostanzialmente ereditiamo dalla legge Stammati di oltre trent'anni fa, perché adesso, obiettivamente, abbiamo un meccanismo troppo incentrato sulla spesa storica. Tuttavia, il Patto di stabilità di quest'anno, contenuto nel decreto-legge n. 112, in qualche modo, creando quattro categorie di enti cerca di superare il sistema della spesa storica e quindi va in questa direzione. Sicuramente non si vuole intervenire a sciabolate nella materia, ma si tratta di creare una logica

tutti i soggetti che interagiscono nella pubblica amministrazione devono seguire una politica economica coordinata, non si può pensare che anche enti locali o Regioni escano da questo tipo di politica economica. Certo, qualche inconveniente, lo devo dire francamente, deriva dal fatto che, una volta che il Patto di stabilità era andato gradualmente adattandosi alle necessità, si era man mano adattato sino ad arrivare, tre anni fa, a definire un meccanismo che aveva come riferimento il totale della spesa, quindi un meccanismo chiaramente correlabile anche al totale delle entrate e quindi al controllo dei flussi di entrata e di spesa, successivamente questo meccanismo è stato abbandonato e siamo tornati al sistema dei saldi. nazionale dei saldi, come anche il sistema dei saldi europei, può andar bene nella contingenza, nel momento eccezionale, ma non funziona a regime, perché un saldo può essere ragionevole, ma dipende dal livello di spesa; infatti, un saldo anche dell'1 per cento ad un livello di spesa molto elevato può essere comunque un rischio per la finanza pubblica, cosa che non sarebbe un saldo magari doppio a livello di spesa molto più basso. Quindi, i saldi vanno bene nel contingente, ma non come strumento definitivo e la cosa la stiamo soffrendo anche nei rapporti con l'Unione europea per il saldo nazionale. Peraltro, un maggiore problema è derivato dal fatto che dall'anno scorso è partito il sistema misto, per cui ci si riferisce alla competenza per la spesa corrente e alla cassa e alla cassa per la spesa in conto capitale. Cosa è successo? Che si sono decise spese di investimento avendo prima, nel 2007, riferimento al totale della competenza, dopodiché, nell'anno successivo, la cassa è stata più bassa, perché ovviamente l'investimento parte con una dose molto bassa; nel 2009 la regolazione dei flussi di spesa è riferita a un miglioramento rispetto all'anno precedente ed ecco che si crea il problema, perché partiamo dal 2008 con una cassa troppo bassa troppo bassa perché scontava l'avvio delle opere. Questo ha creato l'enorme problema che ci troviamo avanti nel 2009. In Commissione si è cercato di dare una risposta a questo tema, perché sono convinto che gli investimenti degli enti locali siano utili anche in funzione anticongiunturale, in vanno più a pronta cassa in termini rapidi; l'abbiamo cercato di fare però ben conoscendo i limiti nei quali ci muoviamo, che sono quelli di non sfondare il tetto dell'indebitamento pubblico e i saldi di Maastricht. Quindi, l'abbiamo dovuto fare con certe cautele, con un meccanismo che presenta qualche farraginosità, però è l'unico che siamo riusciti a definire senza dover

dichiarazione di voto.

Ritirate le tessere che non corrispondono alla presenza Senatore Gasparri, si calmi. Senatore Gasparri, si calmi. La senatrice Segretario sta facendo la verifica che le è stata chiesta dalla Presidenza.

C'è stata una discussione serena, molto seria e costruttiva.

mi associo alle parole del collega Quagliariello per la scheda del presidente Gasparri, ma credo che costituisse un dovere per il senatore Segretario, a fronte di una disposizione della Presidenza, verificare tutte le schede. Non vi era e non vi è alcun significato politico da attribuire ad un gesto di quel genere. Non credo sia il caso. Prego però la Presidenza, visto che la maggioranza dispone di

La Presidenza aveva chiesto, chiede e chiederà sempre che i senatori siano al proprio posto nel momento in cui si effettuano le votazioni.

efficiente per abbassare il costo della politica. Ricordo infatti che quando ci osservano dalla tribuna o in televisione fare "i pianisti" o non rispettare le regole, il costo della politica aumenta, lo spregio e il dispregio di questo Senato aumentano in modo esponenziale. Chiedo dunque ai colleghi senatori di voler di nuovo sottoscrivere una simile petizione alla Presidenza del Senato, che mi premurerò di far circolare, affinché cessi questo scandalo che avvelena le nostre discussioni. Non è serio quello che avviene, e che avviene in continuazione.

vorrei porre all'attenzione di questa Assemblea un tema tra i più delicati con cui il Paese si sta misurando e con il quale il Parlamento italiano si dovrà ancora confrontare in tempi, ci auguriamo, i più brevi possibili: migliorare la qualità e la velocità dei tempi per la giustizia dei cittadini, come da noi più volte sollecitato. Tutto questo va fatto con sollecitudine, ma con grande serenità. Ciò che è accaduto in questi giorni tra le procure della Repubblica di Salerno e Catanzaro non ha precedenti nella storia, sia pure travagliata, della nostra magistratura, ma non è questa la sede per formulare un sia pure succinto giudizio su quegli avvenimenti. Sarebbe un grave errore, ritengo, perché dei fatti si stanno interessando, nelle sedi competenti, gli organi istituzionalmente preposti a garantire la legalità ed il rispetto delle regole in casi di tale anomalia. Tali organi, in particolare il Consiglio superiore della magistratura, si sono tempestivamente attivati dimostrando di sapere e potere esercitare le funzioni che l'ordinamento loro attribuisce per garantire l'efficienza, l'indipendenza e l'autonomia dell'amministrazione della giustizia e noi confidiamo che sapranno, in tempi ragionevoli, fornire le risposte più adeguate al caso. Questo intervento ha, ha, come ho già anticipato, un altro obbiettivo. I fatti di questi giorni hanno generato un senso diffuso di incredulità e al contempo timore di una riforma strumentale della giustizia fatta per colpire autonomia e indipendenza della magistratura,

che i rapporti tra politica, intesa nel suo complesso, e magistratura siano divenuti sempre più difficili negli ultimi anni e che da questo deriva per il Paese uno stato di disagio e di sofferenza, che è nostro compito cercare di rimuovere o alleviare in tempi brevi. Tuttavia, intendiamo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, invitare tutti noi ad una riflessione più attenta, serena e complessiva dello stato della giustizia nel Paese, al fine di ricercare necessariamente, in modo condiviso (questo è l'auspicio), interventi normativi utili per favorire un esercizio della giurisdizione tale da garantire un efficace, tempestivo e corretto servizio della giustizia. Da inizio legislatura ad oggi, di tante auspicate riforme abbiamo assistito solo ad interventi non sistematici e peraltro disorganici. Sarebbe, quindi, un gravissimo errore strumentalizzare un fatto di cronaca come quello per imporre una riforma della giustizia che abbia il sapore di una resa dei conti e di un tentativo di disciplinamento delle funzioni giudiziarie, in particolare di quelle requirenti. Si deve invece ripartire da un'analisi obiettiva e serena delle patologie del sistema giudiziario, non trascurando il profilo centrale dell'inammissibile carenza di risorse destinate alla giustizia, che aggravano quello che è uno dei problemi principali del sistema giudiziario: l'inefficienza, dovuta in primo luogo all'assenza di mezzi e strutture adeguati. Ed a questo va posto rimedio con riforme adeguate e non incidendo sull'obbligatorietà dell'azione penale, sancita dalla Costituzione, e sull'autonomia della magistratura, intesa non come privilegio dei magistrati, ma come garanzia di uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia. Il principio di indipendenza, autonomia e soggezione soltanto alla legge rappresenta difatti badate - un confine invalicabile: solo una magistratura indipendente è garanzia di un'applicazione egalitaria, equa, corretta della legge, idonea ad evitare abusi o disparità di trattamento. E una riforma della giustizia che voglia essere equa, costituzionalmente orientata...

Per fare questo sarà necessario che vengano al più presto discussi in Commissione giustizia i disegni di legge tesi alla riforma dei codici e alla funzionalità degli uffici giudiziari. In attesa e prima che ciò si e prima che ciò si verifichi, proponiamo che questa Assemblea approvi un messaggio di solidarietà e fiducia verso la maggior parte dei magistrati italiani, che quotidianamente, in contesti operativi tutt'altro che agevoli, difendono, nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni, la legalità gravemente e diffusamente violata, ribadendo nel contempo che il Senato della Repubblica

aprire un nuovo dialogo e creare un clima nuovo nell'ambito del quale potranno essere affrontate tempestivamente le riforme che tutti

appoggio la richiesta del collega e considero il momento in cui intervengo la prova provata dell'inaccettabilità dell'idea di rinviare alla fine della seduta gli interventi sull'ordine dei lavori, perché in questo modo essi assumono un significato soltanto formale. Intervengo perché sono costretto a segnalare che oggi pomeriggio, in modo conclamato, si riunirà la pseudo-Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui Presidente, scelto dalla maggioranza dopo 45 volte in cui essa aveva fatto mancare il numero legale, quale unico componente dell'opposizione che ha accettato questa manovra, ha dichiarato che aprirà un'istruttoria sulla trasmissione televisiva Credo che siamo in una situazione ormai grottesca: il Presidente del Consiglio ha il pieno possesso delle comunicazioni di tipo privato; ha il controllo, tramite il Governo, delle comunicazioni di tipo pubblico e noi dobbiamo discutere nella pseudo-Commissione di vigilanza per sindacare l'operato di una trasmissione che "si permette" di avere "uno squilibrio" nella presenza dei politici attuali. Uno squilibrio, capite? L'Aula dovrebbe cogliere questa sfumatura. Nella televisione italiana c'è squilibrio tra la presenza di politici di centrodestra e politici di centrosinistra. Cosa vogliamo, che il centrodestra abbia il totale monopolio della presenza politica all'interno dei mezzi di comunicazione? Vogliamo chiudere qualsiasi tipo di programma in cui non si cantano le lodi del Presidente del Consiglio dei ministri? Dobbiamo assistere a questa scena assurda per cui il Presidente del Consiglio considera se stesso un'istituzione? Egli ha infatti protestato con il Presidente della Repubblica dicendo che se prendono in giro lui prendono in giro l'istituzione. Al Presidente del Consiglio manca l'ABC del pensiero costituzionale, confonde la propria persona fisica con il ruolo: è un gravissimo errore filosofico e istituzionale. Sull'aspetto che ora criticava il senatore Pardi e invece difendeva il senatore Di Giovan Paolo, cioè che le questioni attinenti all'ordine dei lavori, salvo eccezioni, si pongano a fine seduta, difendo